tribuna. (Applausi). Seguito della discussione del disegno di legge: (1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita` nonche´ in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati)

L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonche´ ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

ordine del giorno: I. Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita` nonche´ in materia di processo civile

Colleghi, vi prego di prendere posto e di fare silenzio, perche´ non si puolavorare cosı.

Come ha ricordato il Presidente, esso riguarda la semplificazione, la competitivita e la materia del processo civile. Immagino che, almeno nelle intenzioni di chi ha scritto questo disegno di legge, la semplificazione dovrebbe riguardare anche, se non soprattutto, il processo civile.

l’ammissibilitadel ricorso, ora prevista (in positivo) nei soli casi di decisioni rese all’esito dell’applicazione di principi di diritto in senso difforme da precedenti pronunce della Corte; ricorsi inerenti questioni nuove o sulle quali la Corte ritenga di pronunziarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero in presenza di contrasti nella giurisprudenza della Corte; ove appaia fondata una violazione dei principi regolatori del corretto processo; nonche´ in presenza dei presupposti per la decisione su conflitti di giurisdizione. Ora, pur essendo condivisibile – e noi siamo perfettamente d’accordo – l’esigenza di deflazionare il contenzioso della Corte al fine di valorizzarne la funzione nomofilattica richiamata peraltro dalla stessa Consulta con sentenza recente, n. 170 del 2008, la norma a nostro giudizio

Giacolpisce pensare ad un giudizio costruito in termini di ammissibilita, anziche´ di inammissibilita; e, ancora di piu, colpisce il fatto che in questo modo verrebbe ricondotto nella categoria dell’ammissibilitao inammissibilita

In particolare, poi, suscita perplessita l’esclusiva valorizzazione del precedente giurisprudenziale di legittimitaai fini del giudizio di ammissibilita del ricorso,

modificato di recente, non chiarendo infatti il rapporto tra nuova «inammissibilita» e gia prevista manifesta infondatezza. Dalla formulazione della disposizione sembrerebbe peraltro essere prefigurato un carattere vincolante dei precedenti della Corte di cassazione rimesso alla valutazione della stessa. Ma simili strappi sul terreno delle categorie concettuali e dei principi del corretto processo appaiono ancora piugravi quando si consideri che ad essi si accompagna il rischio di alterazioni profonde sul piano sostanziale della tutela e su quello del ruolo istituzionale della Corte. I margini di opinabilita e discrezionalitainsiti nella identificazione di cio che puoconsiderarsi deciso in modo «conforme» o «difforme» da precedenti decisioni della Corte, di cio che puoritenersi profilo «nuovo» o semplicemente riedizione di tesi gia esaminate in altro giudizio, dei criteri che possono indurre in un caso ad approfondire e in un altro a decidere di non farlo, dei parametri in base ai quali puoritenersi fondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo devono indurre a meditati approfondimenti prima di introdurre formule che l’esperienza potrebbe poi consigliare di abbandonare. E cio tanto piuin considerazione dei dubbi la formulazione del testo apre sullo stesso piano procedimentale, non essendo tra l’altro chiaro in che modo e in base a quali criteri debba essere costituito il collegio cui e devoluto il vaglio di ammissibilita: se tale collegio (peraltro composto inopinatamente da tre magistrati e non da cinque, secondo le regole del collegio di Cassazione) debba essere incardinato all’interno di ciascuna sezione o «a valle» di esse; se il giudizio di ammissibilita sia vincolante per il collegio che decideranel merito il ricorso, essendo comunque da ritenere che la dichiarazione di ammissibilita sotto i profili indicati nell’articolo 360-bis del codice di procedura civile non sia e possa essere di ostacolo alla dichiarazione di inammissibilita, da parte del collegio «ordinario» per profili diversi, cosı come eben possibile che la sentenza impugnata contenga infatti piu statuizioni, alcune soltanto da ritenere ricorribili in base al nuovo testo, profilandosi anche per questa via uno sdoppiamento e una moltiplicazione di tempi e di «passaggi» di giudizi che eesattamente l’opposto di cio di cui ha bisogno la Cassazione. A questo proposito, non so se la maggioranza, nell’appropinquarsi a varare questo testo, ea conoscenza del fatto che presso la Corte di cassazione e giaoperativo un particolare meccanismo,

Resoconto stenografico 3 marzo 2009 del rito camerale, nonche´ di quelli seriali. Essa eaggregata alle sezioni civili ed e composta da un presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a quello necessario per formare un collegio giudicante secondo le norme vigenti. I ricorsi provenienti dalla cancelleria centrale della Corte e destinati ad essere trattati dalle sezioni semplici sono esaminati, in prima battuta, dalla struttura, all’interno della quale sono individuati quelli che possono ovvero devono essere decisi con il rito della camera di consiglio. In tal modo, dunque, si eintrodotto nell’ordinamento della Cassazione – e di fatto e giaoperante – un sistema efficace di selezione dei ricorsi, sul modello di quello francese, che, tuttavia, non risulta essere stato affatto valutato e considerato dal legislatore, o dalla maggioranza di questo istituto

che avrebbe dovuto indurre il Governo e la sua maggioranza a soprassedere, non fermandosi, ma cercando, insieme alla magistratura, all’avvocatura e all’opposizione, soluzioni piuadeguate. Al di la di questi rilievi, va comunque posto in risalto che, se il fine perseguito equello di ridurre la durata del ricorso per Cassazione, deflazionando ad un tempo il carico del contenzioso pendente dinanzi alla Suprema corte, questa norma – lo ripeto e lo sottolineo – edel tutto inefficace, se non addirittura controproducente. Infatti, per i ricorsi dichiarati ammissibili il vaglio giudiziale si raddoppia: l’ordinario giudizio sulla fondatezza o meno sara infatti preceduto da una delibazione preliminare in ordine alla ammissibilitadel ricorso. E[] evidente che questa duplicazione di giudizi non puoche estendere i tempi di decisione del ricorso, aggravando la mole del contenzioso pendente dinanzi alla Corte. Altro che semplificazione; altro che riduzione di termini; altro che dichiarazioni fatte dal ministro Alfano di voler ridurre i tempi del processo. Ne´ del resto potrebbe sostenersi che la preventiva delibazione, da parte del collegio dei tre giudici, in ordine all’ammissibilita del ricorso, possa in alcun modo agevolare il lavoro della sezione in sede di vaglio sulla fondatezza della causa, dal momento che il giudizio preliminare di delibazione attiene ad un profilo assolutamente distinto da quello inerente la fondatezza della causa. Nel caso invece di ricorso inammissibile, per espresso disposto normativo, la relazione conclusiva – badate, questa eun’altra perla di cio che state per varare della fase di delibazione preliminare deve essere notificata alle parti e al pubblico ministero affinche´ possano presentare memorie con le quali contestare o sostenere le conclusioni del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis disegno di legge). Ora, eevidente che tale ulteriore fase di contraddittorio tra le parti non puo che estendere ulteriormente la durata del ricorso e complicare la vita, l’attivitae la produttivita della Corte di cassazione.

in relazione al processo civile in maniera completa ed una delle fasi piuimportanti dell’intero processo civile e quella esecutiva,

il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, quindi situazioni giuridiche particolarmente delicate perche´ riguardano terze persone.

l’emendamento 30.1 riguarda ancora la parte relativa alla fase esecutiva del processo civile e, in particolare, l’inserimento dell’articolo 614-bis che concerne l’attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare.

ottenendo cosı una ingiustificata esclusione delle fattispecie di condanna a favore del lavoratore. Noi siamo convinti e riteniamo convintamente che le cause di lavoro meriterebbe d’esser tutelate e presidiate piudi altre cause; quindi, proprio per questo motivo riteniamo incomprensibile

siamo convinti – che ci possa essere un ripensamento o una migliore valutazione da parte dei relatori e del Governo in proposito, per venire incontro a situazioni particolarmente delicate come quelle relative ai

sia opportuno trasformare l’emendamento 31.4 (testo 2) in ordine del giorno, trattandosi di una materia molto importante che riguarda l’affidamento dei figli in caso di genitori separati.

Il Senato approva.

In particolare con questa norma, visto che estata approvata quella sul calendario del processo, prevediamo che il giudice comunichi tempestivamente al capo dell’ufficio le ragioni per le quali la causa non e stata definita nei termini nei termini previsti dal calendario del processo. Se crediamo nella necessitadi accelerare i tempi del processo, quello civile in questo caso, se crediamo che questo sia un principio sacrosanto che deve essere tutelato,

come scriviamo poi nell’emendamento 33.301, rispetti in maniera assoluta i termini processuali e sia responsabilizzato in questo senso. Quindi, nel caso in cui il giudice non riuscisse a seguire

Grazie,

io confido che qualche valutazione su queste esigenze che, come Partito Democratico, segnaliamo debba essere fatta dai relatori, ma anche dal Governo.

33.301, invito al ritiro, ma, se il senatore Casson lo desidera, noi saremmo pronti ad accogliere un ordine del giorno

del Governo e` conforme al relatore.

non voglio essere offensivo, ci mancherebbe altro! – mi sembra un po’ acqua fresca. Con l’emendamento chiediamo che i giudici rispettino i termini previsti dal codice di procedura civile,

pregiudizialmente contraria a questo emendamento che, fissando tempi certi – come vorremmo tutti – alla durata del processo, imprime al sistema giudiziario efficienza, in nome di un principio di civilta giuridica.

la giustizia civile a livelli di efficienza degni di un Paese industrializzato, di ridare mobilitae respiro ad un sistema

Sono presenti in tribuna a seguire i nostri lavori gli studenti dell’Istituto tecnico per geometri «Filippo Brunelleschi» di Frosinone.

presentato in Commissione, attraverso il quale dovrebbe regolarsi una delle materie piu complesse della procedura civile, ossia la semplificazione e la riduzione dei riti. Uno degli argomenti ricorrenti, quando si parla della malattia del processo civile, e` proprio quello di ricordare che nel nostro Paese esistono 26 o 27 riti. Questa materia era sfuggita al Governo pur essendo presente in tutte le analisi della malattia del processo; un Governo attento aveva perodimenticato di intervenire proprio sul punto:

interventi sotto forma di decreti legislativi da emanarsi entro 24 mesi. ]esattamente il contrario di quella celerita` che si chiede alla giustizia civile quale condizione per lo sviluppo del Paese, perche´ per procedere alla modifica, alla semplificazione, alla riduzione o all’unificazione dei riti

si puo delegare indicando princıpi e criteri direttivi. Abbiamo invece una genericita di formulazione,

le eccezioni di rito e di merito; l’indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova: tutti questi elementi non sono indicati nella delega, eppure attengono alla domanda introduttiva. Cioche poi lascia sconcertati e il fatto che nella delega chiesta dal Governo si chiede di prevedere, nell’ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l’eventuale abrogazione del rito previsto.

questo sia esattamente il contrario del principio sancito dall’articolo 76: si chiede infatti al Parlamento di delegare il Governo ad emanare un provvedimento con cui esso decidera se fare o non fare una cosa, senza che il Parlamento stabilisca in quali condizioni e con quali limiti puofarlo.

inoltre, altri disegni di legge dell’opposizione e della maggioranza sulla materia. Facciamolo dunque seriamente, e non attraverso una norma che sposta i tempi di due anni e con questi contenuti.

Questa norma eun po’ strabiliante per le ragioni gia ricordate dal senatore Li Gotti e, soprattutto, perche´ di questa materia, l’unificazione dei riti, si parla da anni in tutti gli ambienti che hanno a cuore le sorti del processo civile. di una delle questioni fondamentali della riforma del processo civile; non a caso, nei disegni di legge presentati in Senato, da noi come Partito Democratico ma anche da altri senatori dell’opposizione, questo era uno dei principali temi affrontati. Da tutti gli ambienti degli operatori del diritto, per la parte civile (quindi da parte degli avvocati e dei magistrati), si richiedeva di intervenire in questa materia estremamente dispersiva, perche´

da parte del Governo. Con l’articolo 34-bis, relativo alla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, si mette da parte per almeno due anni una riforma che invece sarebbe urgente e qualificante introdurre subito.

sıapplica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennita comunque denominati

E[]questa la sua funzione. Ove tutti i crediti vengano soddisfatti, si realizzerebbe, secondo l’emendamento, una condizione di non punibilita per l’eventuale reato di bancarotta fraudolenta. In buona sostanza, si realizza una condizione premiale. Vorrei rammentare all’Aula che la cultura della premialitaha informato di se´ il processo penale per una lunga stagione e per vicende molto piu gravi e complesse di quelle di cui stiamo oggi discutendo. Credo che il ravvedimento reale di un debitore fallito sia proprio quello di porre in condizione tutti i creditori di ottenere quello a cui hanno diritto, quindi il risarcimento totale del danno, inteso come ravvedimento post delictum e come condizione per evitare la punibilitanel delitto di bancarotta fraudolenta o bancarotta preferenziale, ferme restando tutte le sanzioni che afferiscono ai diritti civili e che sono connesse alla posizione di fallito. Ritengo che il Senato possa esaminare nell’ottica piu giusta e coerente questa proposta, che non intende assolutamente salvare nessuno che non abbia fatto il suo dovere fino in fondo e non abbia estinto tutti i crediti. Confido quindi che il Senato voglia esaminare con attenzione, impegno e rigore questo emendamento, che risponde ad un’esigenza sostanziale, cioequella di far sı

un invito al ritiro.

Partendo da quel testo avevamo predisposto delle norme specifiche molto diverse e piuconcrete. Prendiamo dunque atto della scelta governativa di posticipare nel tempo la soluzione di problemi

che preveda l’integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione… i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili». Qui si tratta del reato di bancarotta fraudolenta, per distrazione, bancarotta documentale, che etipicamente un reato plurioffensivo, che riguarda, cioe, non soltanto l’interesse del singolo creditore ma anche la tutela del commercio nel suo insieme e dell’attivitaimprenditoriale. Consentire in questo modo che si chiudano completamente tutti i reati di natura fallimentare che riguardano una bancarotta, appunto, documentale o sostanziale o per distrazione, crediamo che avvicinerebbe questa norma e questa decisione eventuale del Senato ad un indulto mascherato.

varrebbe per qualsiasi caso di bancarotta e di bancarottiere. A questa forma di indulto mascherato non possiamo dare il nostro assenso. LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

nella materia dei reati fallimentari.

non superare: nella legge fallimentare esiste gial’articolo 241, ossia la riabilitazione nel caso dell’ipotesi di bancarotta semplice. Allora, l’intervento e quindi l’approfondimento sono necessari nell’ambito dell’articolo 241 che prevede proprio l’ipotesi della riabilitazione per il ravvedimento operoso, non disancorandolo dal resto. dal resto. Non capisco francamente la ragione per cui si preveda il ravvedimento operoso per l’articolo 217, quindi la bancarotta preferenziale,

perole norme indicate sono queste. Per quale motivo non prevedere la figura dell’institore, le condotte dell’institore o anche i reati connessi ai falsi per l’accesso al concordato? Tutta la materia dei reati fallimentari puo essere affrontata. Mi rendo conto che l’istituto del ravvedimento operoso operoso esiste nel nostro sistema e quindi puoessere apprezzato. E[ ]ovvio che, se dovesse apprezzarsi per i reati contro il patrimonio, il ladro che restituisce la refurtiva potrebbe chiedere

Invece i ravvedimenti operosi sono previsti come ipotesi attenuatrici di responsabilita e non come scriminanti. Tuttavia, puoaffrontarsi il tema, ma e piuampio di com’e formulato. Esistono degli altri disegni di legge che riguardano la materia fallimentare. La possibilitadi esaminare in un altro contenitore che e giapendente in Commissione giustizia questa materia ritengo che sia la soluzione migliore, perche´ cosı com’eformulato l’articolo e monco, oltre a contenere degli errori che porterebbero a delle incomprensioni,

possa coltivare questa strada nell’ambito dei disegni di legge pendenti.

il decreto-legge n. 185 del 2008 si e modificato questo articolo del codice civile in quanto si eprovveduto all’abrogazione e alla cancellazione del libro soci, libro sul quale si effettuava la pubblicita della titolaritadelle quote e sul quale si poteva contare per stabilire, al momento di compiere una qualsiasi operazione sociale, chi fosse il socio che avesse diritto – ad esempio distribuzione degli utili, convocazione di assemblee; atti, quindi, estremamente rilevanti per la vita di una societa.

dall’iscrizione dell’atto. Tale iscrizione si verifica con l’aggiornamento degli archivi e con la conoscibilita per tutti, compresi gli amministratori di cui dicevo prima, della effettiva titolaritadella quota. L’estensore della norma ha collegato la pubblicita all’atto di deposito del trasferimento della quota; tra il momento del deposito e l’iscrizione, pero, passa un lasso di tempo e il deposito, quindi, e un atto non conoscibile dai terzi che accedono agli archivi informatici.

anche oggi, a chi gestisce il registro delle imprese, ai professionisti e alle imprese stesse, grossi problemi di tenuta del sistema.

numero di anni, si volesse nuovamente modificare il contenuto di questa norma si dovrebbe ricorrere ad una disposizione legislativa invece che ad una disposizione regolamentare, che e nella piena disponibilitadel Governo. Invito dunque il Governo ad utilizzare

dell’adozione di un provvedimento similare, in modo che la modifica introdotta all’articolo 44 possa diventare efficace ed efficiente nel piu` breve tempo possibile.

vecchie tempistiche, quelle piu ampie. Al momento non ci troviamo in condizione di accettare queste riduzioni di tempi, che vanno in senso contrario a quanto giaapprovato. Vorrei,

Grazie,

che mirano sostanzialmente – mi rivolgo soprattutto al Governo – a ridurre un sistema sanzionatorio che, cosı come previsto dall’articolo 50 della finanziaria del 2003, appare in tutta evidenza vessatorio per la sua imponenza e invadenza. Peraltro, atteso il riscontro estremamente positivo positivo registrato a seguito di appositi approfondimenti anche con la Sogei, che gestisce questa quantitaenorme di informazioni che consentono il costante monitoraggio della spesa farmaceutica, credo che i soggetti che consentono questo tipo di

l’osservazione che fu presentata e chiese ai proponenti la trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno di impegno per il Governo.

per trovare una soluzione idonea. Siccome sono convinto che sarebbe una reiterazione dell’impegno gia assunto in questa sede dal Governo, desidero essere rassicurato in tal senso e, a fronte di un’assicurazione di tal fatta, sono assolutamente disponibile al ritiro dell’emendamento 9.0.9.

che consentira di predisporre decreti legislativi sulla quasi totalitadella normativa ambientale. pronunciarsi sull’ammissibilita dell’articolo 9-bis che, a norma dell’articolo 126-bis del nostro Regolamento, edavvero palesemente estraneo all’oggetto del collegato alla finanziaria che stiamo discutendo. Questa estraneita, peraltro, ecertificata dal fatto che sul provvedimento n. 1082 la Commissione ambiente non e stata chiamata a formulare alcun parere, il che dimostra che

Questo articolo estato votato in Commissione senza che ci fosse da parte di alcuno la richiesta di considerare della materia. Osservo inoltre che la materia ambientale, come precedentemente estato detto, e stata affrontata, ad esempio, con riguardo alla semplificazione delle procedure, di cui all’articolo

diversi emendamenti che sembrerebbero testimoniare la coerenza del testo con l’insieme del provvedimento.

della delega ambientale e dei provvedimenti in materia di ambiente e di amministrazione. Quindi, non si puoverificare nessuna fattispecie – questo ovviamente a sommesso avviso del Governo – di differenziazione di materia rispetto al contenuto originario del provvedimento ne´ di materia nuova rispetto a quello che era previsto nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Sotto questo profilo, quindi, mi risulterebbe difficile ritenere che l’articolo 9-bis sia una norma

nel 2002 e che adesso arriveremo al 2011, ci saranno dieci anni di totale incertezza normativa per i cittadini, le imprese e gli operatori che operano in campi assolutamente sensibili, in gran parte dei campi oggetto della legislazione ambientale: si va dalle acque ai rifiuti, dalla valutazione di impatto ambientale alla regolamentazione del danno ambientale fino ai temi legati all’inquinamento dell’aria. Oltretutto, l’articolo 9-bis rende ancora meno rilevante e meno cogente il controllo esercitato dal Parlamento: mentre infatti nella prima legge delega del 2004 veniva previsto un doppio passaggio nelle Commissioni parlamentari competenti per gli schemi di decreti legislativi, in questo caso il passaggio diventa uno solo.

e questo credo dovrebbe accrescere le preoccupazioni, non solo dell’opposizione ma di tutto il Senato e di tutto il Parlamento rispetto alle conseguenze che questo articolo 9-bis rischia di produrre in termini di incertezza normativa e anche nel merito. Inoltre, si richiamano in modo generico gli indirizzi previsti dalla legge delega del 2004; sono passati cinque anni, molti dei temi che hanno a che fare con i grandi capitoli dei decreti legislativi che verranno predisposti hanno naturalmente mutato le loro caratteristiche. davvero che dal punto di vista della dialettica tra Governo e Parlamento, e anche del merito, questo articolo 9-bis aggiunto in questo collegato alla finanziaria sia un errore molto grave da parte del Governo e, se verra` approvato, da parte della maggioranza di questa Aula.

Signor Presidente, faccio presente che l’emendamento in questione potrebbe teoricamente avere degli effetti contrari rispetto alle direttive comunitarie vigenti e creare delle discriminazioni nelle procedure di gara.

salvo il contenuto proprio dell’emendamento, cioeil riferimento alla possibilita di istituire altri tipi di indirizzi di posta elettronica certificata, omettendo pero` la parte che era stata dichiarata inammissibile.

che rischiano di essere tagliate fuori da un determinato circuito di lavori, con conseguenze sociali ed economiche cospicue. Anche in questo caso, mi sono modestamente fatto carico di un problema relativo alle tecnologie telematiche delle comunicazioni, per istanze che vengono dall’azienda postale, che si vuole mettere nella condizione di offrire un servizio piuefficiente, ma al tempo stesso certificato ed affidabile a tutti gli effetti, nazionali ed internazionali,

sparirebbe la lettera a) del testo originario da me proposto, mentre si integrerebbe il punto b), e diventerebbe il numero 1) quello che era numero 2) nel testo di partenza. Ora l’integrazione che propongono il Governo e il relatore

quale tipo di difficolta applicative, quale tipo di aggravio economico esistono? Se mi si spiega cioe mi si convince non ho difficolta ad accettare integralmente la riformulazione che viene proposta,

riesce a dare un grosso contributo a tutte le amministrazioni comunali. In questo particolare periodo in cui il settore ambientale edi notevole rilievo e nell’interesse di tutti si riescono a produrre 200 chilowatt di energia elettrica

dal Governo. E[` ]approvato. Nella seduta antimeridiana di oggi la Presidenza ha informato l’Assemblea di aver trasmesso nuovamente l’articolo 26-quater alla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento. Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

2-quater, del Regolamento – sentito il rappresentante del Governo – osserva che la norma eomogenea, nel suo contenuto e nelle sue finalita complessive, rispetto alle materie indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 e nella relativa risoluzione nell’ambito delle politiche per la semplificazione e per la competitivita`». PRESIDENTE. Alla luce del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, la Presidenza conferma l’ammissibilita` dell’articolo 26-quater. LUSI (PD).

Non devo ricordare il fatto che stiamo trattando di un collegato alla legge finanziaria e che, per quanto riguarda le materie in esso trattate, queste si trovano all’interno del combinato disposto, per quanto riguarda questo esercizio, del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica 2009-2013, e, signor Presidente, della Nota di aggiornamento allo stesso Documento che estata approvata successivamente.

Presidente, il tema trattato dall’articolo 26-quater riguarda la revisione, attraverso un procedimento di legge delega, di alcune questioni rimaste delicatamente in sospeso nel nostro ordinamento, perche´ non risolte, relative al processo amministrativo. marzo 2009 trattando del procedimento amministrativo, stiamo trattando del processo amministrativo e in questo senso io non devo spiegare a nessuno quale sia la differenza, essendo tutti amabilmente piuesperti del sottoscritto. del dibattito che si e svolto in materia, ha precisato in piudi un’occasione che i termini del processo amministrativo non sono affatto inclusi ne´ nel Documento di programmazione economico-finanziaria ne´ tantomeno nella Nota di aggiornamento Non v’e chi non veda, signor Presidente, che l’ammissibilitadell’articolo 26-quater e totalmente al di fuori della linea di ammissione tematica prevista nei temi del Documento di programmazione economico-finanziaria. visionare la pagina 14 del Documento di programmazione economico-finanziaria e la Nota di aggiornamento a pagina 7, ella trovera, signor Presidente, sia le questioni che riguardano il procedimento amministrativo (nella prima) sia le materie del processo civile (nella seconda).

legge delega relativa al processo amministrativo sia possibile perche´ nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria si tratta del processo civile. Fino a prova contraria le questioni che riguardano il diritto civile ineriscono ai diritti soggettivi e, fino a prova contraria, le questioni che riguardano il diritto amministrativo e il processo amministrativo riguardano gli interessi legittimi. Non sta nemmeno in piedi la giustificazione secondo la quale alcune fasi del procedimento di rito, quello relativo, nel caso, del codice di procedura civile, vengano utilizzate all’interno del processo amministrativo. Lei, Presidente, sa meglio di me, sia per l’esperienza professionale che la contraddistingue, sia per quella di gran lunga piuistituzionale che le due questioni sono assolutamente distinte e distanti. Vertendo in materia di collegato alla finanziaria, non siamo idonei a trattare la materia del processo amministrativo con una norma delega inserita dentro un collegato il cui tema non sia stato indicato a monte ne´ nel Documento di programmazione economico-finanziaria, tantomeno nella Nota di aggiornamento. Quindi, signor Presidente, ben conoscendo che i termini regolamentari danno alla sua dichiarazione una sorta di inemendabilita, la invito fortemente, a nome dei colleghi del Gruppo del Partito Democratico, a vedere

le materie del procedimento amministrativo relativo alla semplificazione e all’incentivazione allo sviluppo e, nel secondo, le questioni che riguardano il processo civile. In nessuno dei due, ne´ nel DPEF, ne´ nella Nota di aggiornamento allo stesso, ella trovera questioni che riguardano il processo amministrativo.

e perche´, come Presidente di una delle due Commissioni che hanno portato in Aula questo provvedimento… PRESIDENTE.

Lo darorapidamente. Faccio due sole osservazioni. In primo luogo, la questione di cui stiamo discutendo e stata posta in Aula per la prima volta nella scorsa seduta. Faccio presente che le norme di cui stiamo parlando sono state presentate al Senato il 19 novembre 2008. A questa proposta i senatori dell’opposizione hanno presentato 28 emendamenti, 18 dei quali sono stati approvati e due assorbiti; tutto questo nel lavoro delle Commissioni. Dopo essere entrati nel merito e dopo che sono stati accolti i 18 emendamenti, hanno posto in Aula il problema dell’inammissibilita. di programmazione economico-finanziaria, quando si parla di trasparenza della pubblica amministrazione e di semplificazione, e evidente che nessuno puopensare di cambiare le regole della pubblica amministrazione e non lo strumento processuale. Concludo peraltro, rispondendo alle osservazioni del senatore Lusi sul problema di connessione tra la giustizia civile e la giustizia amministrativa, leggendo una lettera che il 9 gennaio 2008 l’allora presidente del Senato Franco Marini invio ai Presidenti della 1ª e della 2ª Commissione risolvendo una questione di competenza, rilevando l’esigenza – leggo testualmente «di prendere atto dei piurecenti sviluppi legislativi in materia, orientati a forme di tutela piu simili a quelle della giustizia civile. In particolare, la legge n. 205 del 2000, che ha attribuito al giudice amministrativo ambiti di giurisdizione e strumenti di tutela assai piupenetranti che in passato, ad esempio riconoscendo al privato la possibilita di agire in giudizio non solo per fini meramente impugnatori, ma anche per il riconoscimento dei diritti patrimoniali conseguenziali»; sin qui il presidente Marini. Qui mi fermo per sostenere che la decisione della Commissione bilancio e la conseguente decisione della Presidenza sono assolutamente in linea con lo svolgimento dei fatti e con situazioni gia` precedentemente affrontate dalla Presidenza del Senato.

senatore Casson, Grazie, sul modo di procedere da parte del Governo con questa legge delega. Va peraltro riconosciuto che i princıpi e il contenuto di alcune norme che sono indicate sarebbero proprio quelli che dovevano essere contenuti nelle norme all’interno di un disegno di legge completo di riforma del processo amministrativo. Ricordo soltanto alcuni di questi punti perche´ e bene che essi rimangano agli atti. Sicuramente merita apprezzamento la scelta di introdurre norme volte alla razionalizzazione e alla riduzione dei tempi dei processi, garantendo contemporaneamente il rigoroso rispetto dei diritti e delle garanzie inviolabili della difesa. Noi condividiamo anche la proposta di riordinare i casi di giurisdizione estesa al merito, soprattutto perche´ in questa sede epossibile garantire la dovuta tutela anche ai cosiddetti interessi amministrativamente protetti. ]inoltre condivisibile la scelta di prevedere dei rimedi dichiarativi, costitutivi di condanna e idonei a soddisfare la parte vittoriosa. Si condivide poi la proposta di generalizzare la tutela ante causam, come auspicato dalla Corte di giustizia europea, giaprevista dalla disciplina degli appalti, soprattutto se concepita attenuando il vincolo di strumentalita dell’azione cautelare rispetto alla fase cognitoria. Ora, noi avremmo preferito che tutte queste considerazioni e il contenuto di queste norme fosse trasfuso in una legge immediatamente operante e che gli operatori del diritto avessero da subito potuto utilizzarla nel corso della loro attivita. Cosı non estato e ancora una volta, come abbiamo gia avuto modo di sottolineare, in materia di conciliazione, di diritto commerciale, commerciale, di processo esecutivo e di ragionevole durata dei processi civili, il Governo rinvia di anni delle soluzioni che potevano essere adottate in fretta.

all’entrata in vigore, dopo la ratifica odierna, avvenuta sulla base di un dibattito durato pochi minuti in sede di Parlamento (con rispetto parlando) libico, del famoso Trattato Italia-Libia.

quel Paese. Anche grazie alla mobilitazione italiana lanciata da Marco Pannella, fatta propria tanto dalla Camera quanto dal Senato, si e riusciti a far emergere un processo che stava diventando nascosto e che si econcluso, in questo caso, con l’assoluzione (almeno altri due processi sono ancora

2009 situazione che determina, credo per tutti noi, uno stato di particolare disagio nel rapporto con l’opinione pubblica.

i gestori della buvette del Senato ricevono dal Senato stesso un significativo trasferimento compensativo

era possibile individuare lo spazio per una riduzione significativa dei prezzi, E quindi, francamente non so giustificare in nessun modo la decisione dei senatori Questori che, in presenza di una situazione di questo tipo, hanno concluso per il mantenimento del trasferimento compensativo nelle stesse dimensioni di prima, di fatto consentendo la riduzione dei prezzi e in quella proporzione. Penso si tratti di una decisione molto grave e seria nel contesto di crisi drammatica nella quale versa il nostro Paese e che sia noi sia i senatori Questori, signor Presidente, dovremmo tutti trarne spunto per un mutamento radicale di orientamento. applicare una riduzione della quota corrispondente a quella derivante dal mancato introito per riduzione percentuale dei prezzi in riduzione del trasferimento all’impresa da parte del Senato a compensazione del mancato introito. In secondo luogo, dovremmo assumere l’immediata decisione di far praticare prezzi di mercato, signor Presidente, da questa benedetta buvette

voluto immediatamente intervenire con i senatori Questori, piuche altro perche´ non era indifferente a quanto stava accadendo, e ha voluto immediatamente recuperare la situazione cosı come ho appena detto. E[` ]chiaro che fra quattro mesi, a conclusione della gara, avremo certamente un solo gestore, con un abbattimento notevole dei costi che attualmente abbiamo per le quattro aree di ristorazione. (Applausi del

a me sembra un dovere istituzionale. Questa mattina abbiamo dovuto fare una conferenza stampa con l’adesione di 60 parlamentari per rafforzare tale richiesta e mi sembra che sarebbe dovere del Governo dire che cosa pensa.

La seduta e` tolta